L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

delle imprese costrette a sospendere le proprie attività, scongiurando in tal modo il rischio di disastrosi licenziamenti e assicurando, altresì, quel patrimonio di professionalità che poi ha consentito, alle medesime imprese, di essere pronte per la ripresa, attraverso il dispiegamento di ingenti risorse dello Stato. Come emerso anche nelle prime fasi di attuazione di tali misure straordinarie, non sono purtroppo mancati deplorevoli casi di utilizzo improprio, se non addirittura fraudolento, di tali provvidenze. Diverse imprese hanno infatti utilizzato la cassa straordinaria Covid-19 anche senza la contrazione delle attività e hanno addirittura utilizzato la medesima cassa, pur continuando ad impiegare i propri dipendenti, per lo svolgimento ordinario delle proprie prestazioni lavorative. In particolare, secondo quanto riportato da alcuni articoli di stampa e nella recente inchiesta del programma televisivo «Report», tra le imprese che avrebbero impropriamente utilizzato la cassa Covid-19 figurerebbe anche la Visibilia editore, società quotata in borsa e a suo tempo controllata, per il 48,6 per cento, dalla allora senatrice Santanchè, attualmente Ministro. Una *ex* dipendente della società, con ruoli di responsabilità, sarebbe stata posta in cassa integrazione a ore zero a sua insaputa. La Visibilia si sarebbe, quindi, avvalsa delle citate misure straordinarie durante l'emergenza, anche se la dipendente continuava a svolgere il proprio lavoro. L'*ex* responsabile, questa stessa dipendente ha esplicitamente dichiarato di aver continuato a lavorare per la società del ministro Santanchè, per scoprire solo successivamente che la società la pagava attraverso dei rimborsi spesa chilometrici e senza essere mai stata informata di trovarsi in cassa integrazione.

dipendenti. Qualora fossero confermate le vicende ora riportate, esse evidenzierebbero gravi lesioni dei diritti dei lavoratori e un uso illegittimo degli strumenti straordinari messi a disposizione dal Governo. Alla luce di tutto questo e dando seguito all'impegno che proprio il Governo ha preso pochi giorni fa di appurare se vi fossero stati degli illeciti anche da parte di Visibilia e di recuperare le risorse eventualmente erogate impropriamente a Visibilia, le pongo la

attività ispettive del lavoro. Dunque, in quanto tempo pensate di poter rendere note queste informazioni e recuperare eventualmente le risorse che fossero state erogate in maniera illegittima?

sociali*. Signor Presidente, con l'atto di sindacato ispettivo in esame, la senatrice interrogante chiede di conoscere quali iniziative di competenza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare al fine di verificare i comportamenti della società Visibilia Editore SpA in merito alle vicende riportate in questi giorni dagli organi di informazione, e se intenda attivarsi per il recupero di eventuali somme indebitamente percepite. Come ho già avuto modo di riferire ieri alla Camera dei deputati rispondendo a un'analoga interrogazione, segnalo in via preliminare - come è certamente noto all'interrogante - che dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2015 il Ministero non ha poteri ispettivi, che sono stati totalmente trasferiti all'Ispettorato nazionale del lavoro-Agenzia per le ispezioni del lavoro. Nella materia oggetto della presente interrogazione ha poteri di verifica anche l'INPS ai fini della valutazione della legittimità della concessione degli ammortizzatori sociali. Ricordando che su entrambi gli enti il Ministero mantiene esclusivamente poteri e funzioni di vigilanza, si coglie l'occasione fornita da questa interrogazione anche per confermare che è in corso il rafforzamento dell'organico del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro con l'inserimento di circa 800 unità di personale nel corso del 2023, che andranno ad aggiungersi alle circa 5.000 unità già in servizio. L'Ispettorato si avvale anche dell'attività del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, che può contare su circa 450 unità in servizio, nonché - in regime di convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 48 del 2023 - anche della Guardia di finanza. In ordine alla concessione della cassa integrazione guadagni, è bene inoltre ricordare che la normativa vigente - nel caso della cassa Covid, in particolare l'articolo 22-*quater* del decreto legge n. 18 del 2020 - prevede che, nel caso in cui sia provato l'indebito accesso del datore di lavoro all'utilizzo degli strumenti di integrazione salariale, le somme anticipate siano prontamente recuperate con una procedura amministrativa, fatta salva l'eventuale responsabilità penale in caso di commissione di reati connessi alla richiesta di concessione. Fatte queste doverose premesse, si rappresenta alla senatrice interrogante che sulle vicende oggetto della presente interrogazione confermata la piena e costante attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine alle attività svolte e in corso di svolgimento da parte degli organismi ispettivi vigilati, sulle quali sarà possibile fare una piena valutazione soltanto agli esiti delle stesse.

Giorgia Meloni andava gridando che il Governo doveva dare 1.000 euro a tutti con un *click.* Il Governo Conte fece molto di più: fece in modo che la cassa integrazione potesse arrivare subito a qualunque impresa ne facesse richiesta, sulla fiducia. Quindi, fa davvero tremare l'idea che delle imprese, guidate da una donna di Stato quale la Santanchè già era, possano avere approfittato di un tale momento di fragilità del del Paese e piegato dette misure ai propri interessi. Dico di più: la ministra Santanchè, non più di una settimana fa, si è presentata in quest'Aula con la determinazione di mentire. mentire. Infatti, signora Ministra, se lei sapesse che deve venire in Aula a riferire rispetto alla sua situazione penale, penso che si premurerebbe di fare un accesso al certificato pochi giorni prima di venire in Aula. Invece la ministra Santanchè è venuta a sventolare un certificato vecchio di oltre sette mesi, con l'intenzione premeditata di mentire. Siccome la ministra Santanchè proprio oggi ha affermato

Ministro, parliamo di cose serie. A partire dal primo maggio 2023, il territorio dell'Emilia-Romagna è stato tragicamente colpito da eventi alluvionali di gravissima portata, caratterizzati da straripamenti, causando la drammatica perdita di diciassette vite. Nel rendiconto presentato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna al Governo il 15 giugno scorso, la stima provvisoria dei danni ammonterebbe a circa 9 miliardi di euro. L'alluvione ha determinato danni devastanti all'intero tessuto economico e produttivo delle aree colpite, dai settori direttamente coinvolti dagli eventi alluvionali - come l'agricoltura e la filiera alimentare - fino alle migliaia di industrie e imprese del turismo che costituiscono una delle dorsali più produttive e virtuose del nostro sistema Paese. Un'analisi presentata da Unioncamere Emilia-Romagna stima che il valore aggiunto atteso per il 2023 per i Comuni colpiti dall'alluvione ammontasse a circa 40 miliardi di euro e che, a seguito della stessa, si rischia un'incidenza negativa su tale valore compresa tra il 18 e il 26 per cento. Quindi, una prima stima fornita da Confindustria, Il quadro che emerge dai dati testimonia una situazione di grave crisi in territori strategici del nostro sistema economico, che mette a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e rende altresì incerta e difficoltosa l'attività svolta da tantissimi professionisti e lavoratori autonomi.

prevede, all'articolo 7, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali che stabiliscono una procedura per fornire ai lavoratori subordinati dei territori colpiti una integrazione del reddito a carico dell'INPS. Il decreto stesso, all'articolo 8, disciplina una misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi che l'INPS deve riconoscere e attribuire a seguito di apposita domanda. Bene, Ministro, mia domanda è se è possibile valutare fin da ora l'efficacia delle misure adottate per salvaguardare l'occupazione nei territori colpiti dall'alluvione e quale impatto tali misure hanno avuto sul tessuto economico di tali territori. PRESIDENTE. Il ministro

adottati per far fronte all'emergenza che ha colpito lo scorso mese di maggio la Regione Emilia Romagna e alcuni Comuni delle Marche e della Toscana. Con il decreto-legge n. 61 del 2023 sono stati introdotti, tra le altre misure, un ammortizzatore unico per i lavoratori dipendenti del settore privato e per i lavoratori agricoli, nonché un'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi. I due strumenti sono stati concepiti per consentire maggiore celerità e tempestività sia nella procedura di richiesta da parte dei lavoratori interessati sia in quella di erogazione della prestazione da parte dell'INPS. Entrando nel dettaglio delle due misure introdotte dal Governo, rammento che possono fruire dell'ammortizzatore unico, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, i lavoratori dipendenti o agricoli che alla data del primo maggio risiedono, sono domiciliati o lavorano presso un'impresa ha sede legale o operativa in uno dei territori interessati dagli eventi alluvionali, ovvero che siano impossibilitati a recarsi al lavoro in ragione dell'evento straordinario. Inoltre, con riferimento ai lavoratori agricoli, la misura di sostegno è prevista anche in favore di coloro i quali non avevano un rapporto lavorativo alla data dell'evento straordinario emergenziale. Per i lavoratori del settore agricolo la misura di sostegno per le giornate di sospensione delle attività lavorative è equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse. Voglio ribadire che sostenere le aziende e i lavoratori dei territori alluvionati rappresenta una priorità fondamentale per il Governo ed è per questo che abbiamo agito con celerità in un'ottica di semplificazione procedurale, prevedendo il pagamento diretto della misura da parte dell'INPS e la non applicazione dei limiti temporali previsti a legislazione vigente per i trattamenti di integrazione salariale, nonché il venir meno dell'obbligo di versamento del contributo addizionale. Con riferimento all'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi, questa è riconosciuta in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa e gli iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, sempre per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, per un importo pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione per un totale di 3.000 euro. Per rendere tempestiva l'erogazione del sussidio si è individuata anche in questo caso una procedura semplificata gestita dall'INPS. A copertura delle misure sono stati stanziati circa 900 milioni di euro, di cui 253,6 per il sostegno al reddito dei lavoratori autonomi. Voglio informare i senatori interroganti che alla data dell'11 luglio 2023, sulla scorta dei dati forniti da INPS, risultano presentate in totale 24.045 domande, di cui 12.507 relative alla misura *una tantum* destinata ai lavoratori autonomi e 11.538 per l'ammortizzatore unico. I pagamenti avviati alla stessa data risultano in totale 10.036, mentre 9.506 sono i pagamenti già ricevuti dai richiedenti. Questi dati confermano che la semplificazione delle procedure adottata ha consentito di dare una risposta immediata, efficace e tempestiva ai lavoratori e alle aziende. Concludo confermando la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti delle popolazioni colpite dall'alluvione attraverso uno scrupoloso monitoraggio dell'andamento delle misure sopra descritte, valutando la possibilità di rendere strutturale e ordinario l'istituto dell'ammortizzatore unico emergenziale a garanzia di un sostegno immediato e tempestivo a favore delle popolazioni colpite da eventi straordinari.

mettere in risalto la cifra stanziata a copertura delle misure. Si tratta - come lei ha detto - di oltre 874 milioni di euro, di cui 620 milioni per l'ammortizzatore unico per i lavoratori dipendenti e 253 milioni milioni di euro a sostegno del reddito dei lavoratori autonomi. Un'altra misura che reputo assolutamente importante è la procedura semplificata che potrà consentire anche per provvedimenti futuri

che questi siano gli atteggiamenti che devono caratterizzare l'attività del Governo: prontezza rispetto agli eventi straordinari e calamitosi; concretezza delle misure messe in campo; misurazione costante durante l'applicazione del provvedimento dei benefici, in modo da poter mettere in campo rapidamente i necessari correttivi. In questo caso il provvedimento è giusto, appropriato, tempestivo, procede regolarmente e di questo, evidentemente, non posso che dichiararmi soddisfatto. La stessa identica cosa non posso fare per i processi sommari, per la pretesa di rovesciamento dello Stato di diritto, signor e per quello che poco fa abbiamo ascoltato in quest'Aula rispetto ad accadimenti e fatti che sono tutti in capo all'autorità giudiziaria, che avrà modo di giudicare e valutare la rispondenza delle dichiarazioni rese, rispetto ai fatti accaduti. Di questo invece mi dichiaro molto preoccupato perché, quando la politica assume

come sappiamo, il diritto alla salute è sancito nella nostra Costituzione all'articolo 32 ed è un diritto fondamentale, non solo perché riguarda sia la salute dell'individuo che l'interesse della collettività, perché impegna in maniera responsabile il Governo sulle misure da adottare. Sappiamo che il Piano nazionale per il Governo delle liste d'attesa prevede che le Regioni e i Comuni debbano definire i piani locali con la partecipazione dei cittadini, ma la previsione finora, purtroppo, è rimasta di fatto lettera morta. Sappiamo anche che il PNRR, nell'ambito della Missione 6, destina 2 miliardi di euro proprio al potenziamento dell'assistenza sanitaria di prossimità e alla riduzione delle ospedalizzazioni non urgenti, tramite l'attivazione di 1.350 case Sia però sulle liste d'attesa che sulla riforma dell'assistenza territoriale e la sua integrazione con i servizi, anche ospedalieri, già esistenti e non solo, e non solo, gli interventi adottati finora dal Governo, purtroppo, sono stati volti soltanto a tamponare l'emergenza, piuttosto che affrontare le problematiche del Servizio sanitario nazionale in un'ottica di lungo periodo.

emergenza, anche attraverso l'osservatorio nazionale delle liste d'attesa, per renderle più uniformi, chiare e fruibili ai cittadini e soprattutto dando informazioni sui tempi di attesa e sulle modalità di accesso alle cure. Purtroppo, però, come abbiamo visto anche dall'ultimo rapporto di Cittadinanzattiva del 2023, questo non si sta verificando. L'urgenza e l'emergenza le conosciamo bene, le liste d'attesa sono ormai diventate intollerabili in tutte le Regioni del Nord, quali iniziative intende adottare per ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, garantendo piena effettività al diritto alla salute, al fine anche di scoraggiare in ogni modo il fenomeno della rinuncia alle cure. Sappiamo che già oggi il 40 per cento persone rinuncia a fare prevenzione. Chiediamo allora di sapere quali iniziative, di competenza del Ministro, si intendono adottare per risolvere le criticità già da me esposte e anche come garantire piena tutela al fondamentale diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, che oggi sappiamo essere pregiudicato anche dalla carenza di personale sanitario, di medici e infermieri, di farmaci, di strutture e dai tempi di attesa che,

risalenti negli anni, per le quali dall'inizio del mio mandato sto avviando ogni azione di contrasto. È nota la problematica relativa ai lunghi tempi di attesa per il conseguimento di prestazioni sanitarie, diagnosi, interventi terapeutici, assistenziali e riabilitativi che affligge l'Italia, in merito al quale anche il Rapporto civico sulla salute 2023 di Cittadinanzattiva ha fornito un'analisi di sofferenza per i cittadini. A tal riguardo, devo ricordare che la legge di bilancio 2022 ha introdotto specifiche disposizioni e stanziamenti volti al recupero delle prestazioni non erogate per la pandemia. Con l'entrata in vigore, poi, del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022 è stata data la possibilità a Regioni e Province autonome di rendere disponibili per l'equilibrio finanziario 2022 risorse correnti non utilizzate al 31 dicembre 2022 per dare attuazione ai piani operativi regionali per il recupero delle liste d'attesa. Per supportare e monitorare l'azione delle Regioni, il Ministero della salute ha emanato, di conseguenza, con circolare 30 maggio 2023, peculiari indicazioni in conformità a quanto disposto nel summenzionato decreto-legge. In particolare, Regioni e Province autonome che hanno a disposizione un residuo delle risorse correnti non utilizzate al 31 dicembre 2022 possono rendere disponibili queste risorse per le finalità legate a garantire la piena attuazione dei piani operativi regionali per ridurre le liste d'attesa. Le Regioni e le Province autonome che, all'esito delle attività di aggiornamento delle liste consolidamento dei dati trasmessi al Ministero della salute, hanno ancora prestazioni da erogare riferibili alle liste d'attesa generatesi durante il periodo pandemico possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2023. Inoltre, Regioni e Province autonome possono avvalersi fino al 31 dicembre 2023 delle misure specificatamente previste dalla legislazione vigente, che ora ricordo. Per il recupero dei ricoveri ospedalieri, ambulatoriali e di *screening* con queste modalità: prestazioni aggiuntive della dirigenza medica sanitaria veterinaria e professioni sanitarie dipendenti dal Sistema sanitario nazionale con tariffa oraria aumentata; prestazione aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente dal Sistema sanitario nazionale con aumento della tariffa oraria; reclutamento attraverso assunzioni a tempo determinato di personale di comparto e della dirigenza medica sanitaria sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie anche in deroga e vigenti contratti collettivi del lavoro. Insieme al summenzionato atto di indirizzo e altresì chiaro che, per il recupero delle prestazioni ambulatoriali e di *screening*, in parziale alternativa a quanto indicato nei punti precedenti, Regioni e Province autonome possono incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale. Viene acclarato che è consentito il ricorso alle strutture private accreditate in deroga alle limitazioni disposte dalla vigente normativa. Con il medesimo documento di indirizzo è stato previsto il prosieguo delle attività di monitoraggio e supporto fornito alle Regioni e Province autonome da parte del Ministero della salute e di Agenas. Questi sono problemi - come dicevo prima - che derivano da scelte errate e prolungate negli anni che oggi siamo chiamati a fronteggiare. Ne citerò due. La prima è il blocco indiscriminato del *turnover*,

Come detto poc'anzi e come ribadito più volte, abbiamo stanziato fondi straordinari per l'abbattimento delle liste d'attesa e ci attendiamo che tutte le Regioni li sappiano impiegare con urgenza e al meglio. Stiamo lavorando in controtendenza. Vogliamo non più *bonus* e misure tampone o arrotondamenti vari, ma interventi strutturali, con più soldi per il personale medico e sanitario, più tutele per gli operatori sanitari, più fondi per retribuire gli straordinari, più posti per chi vuole studiare medicina.

sono anche molto rammaricata, perché lei si è ostinato a non dare nemmeno un dato del livello di recupero dei *target* dopo il Covid rispetto a tutti i temi delle liste d'attesa. Glieli do io i dati che lei non ha voluto

Solo questi dati le dovrebbero evidenziare che siamo di fronte a un'emergenza di carattere nazionale. Questo Governo può anche continuare a dire che tutti i problemi si sono ereditati dal passato. il problema è che, dopo sette-otto mesi, qualche problema bisognerebbe cominciare a risolvere e purtroppo la situazione in termini di liste d'attesa nel nostro Paese è esplosiva. esplosiva. Che cosa significa? Significa che ci sono delle Regioni nelle quali le persone rinunciano a curarsi. Le faccio un esempio: secondo un articolo uscito ieri un giornale della mia Regione, la Liguria, il 5,8 per cento nel 2022 ha rinunciato alle cure. Questo dato dovrebbe indurci a mettere in atto delle politiche in controtendenza.

che vuole mettere in atto un progetto di autonomia nel nostro Paese. Ma bisogna riscontrare il fatto che non c'è omogeneità in tutta Italia rispetto alle prestazioni di carattere sanitario. Tuttavia, quello che più mi preoccupa è il fatto che non ci sia, nella sua relazione, alcun riferimento rispetto a cosa volete fare, a come volete cambiare questa situazione, al tipo di investimenti che volete mettere in campo sul sistema sanitario e a come ritenete di approcciare

Stimo il suo lavoro e sicuramente non c'è un approccio ideologico da parte nostra. Le devo dire però, Ministro, che la relazione di oggi su un tema così serio, in diretta Rai, senza un dato, senza un riferimento, senza dire cosa volete fare come Governo, è qualcosa che non solo mi sorprende, ma mi rammarica e penso, con me, tutti gli italiani.

Signor Ministro, credo che anche lei sia stato raggiunto dalle stesse lamentele che hanno raggiunto me, da parte dei cittadini, dei lavoratori e delle persone che vorrebbero occuparsi di sanità del Comune di Velletri e di tutti i Castelli. E ricordo che lei è stato recentemente in visita a Velletri, per occuparsi della problematica dell'ospedale Colombo. Non so se poi è riuscito ad andare a vedere anche la situazione dell'istituto di Velletri che fa capo alla proprietà del San Raffaele. Nel 2011 - come forse credo lei sappia - la direzione regionale ha disposto la revoca, per questo ospedale, della sola autorizzazione di cui il presidio risultava titolare. Pertanto veniva - ahimè - chiuso, non senza qualche simbologia purtroppo di natura politica, che nella sanità - a mio parere - non ci dovrebbe mai essere. una chiusura, quella del San Raffaele, che ha pesato come un macigno, vista la situazione al limite della sanità di Velletri - come dicevo poc'anzi - dove anche l'ospedale civico, del quale lei si è occupato, sta subendo da anni drastici ridimensionamenti e si è anche sfiorata la chiusura. La chiusura dei presidi territoriali - come tutti sappiamo nostra sanità, come abbiamo purtroppo visto durante la drammatica pandemia. La struttura sanitaria è stata chiusa per indagini della procura di Velletri, che si sono chiuse con l'assoluzione completa e con formula piena, per insussistenza del fatto, di tutti gli imputati da ogni contestazione a loro ascritta. Persino la Corte dei conti ha sottolineato che non vi era alcuna ipotesi di responsabilità erariale. La struttura è stata chiusa nonostante fosse un fondamentale presidio per la riabilitazione e per reparti importanti di medicina, di chirurgia e di cardiologia. Accertata quindi l'insussistenza del presupposto della revoca, quello che oggi possiamo rilevare è come i cittadini della Regione Lazio si siano visti privati *de facto*, per ben dodici anni, di un presidio attrezzato per lo svolgimento di attività sanitarie. Vista l'idoneità, mi chiedo, signor Ministro, se per caso è a conoscenza della situazione e per quali motivi non si sia ancora proceduti al ripristino dell'autorizzazione all'esercizio dell'accreditamento in favore della struttura di Velletri, che speriamo possa essere riaperta al più presto, perché anche la commissione sanitaria

*ministro della salute*. La questione delineata nell'atto ispettivo in esame rientra negli ambiti di competenza della Regione Lazio, alla quale ho chiesto di relazionarmi compiutamente. Risulta, con determinazione del 22 giugno 2011, che la Regione ha revocato l'autorizzazione all'esercizio alla casa di cura San Raffaele di Velletri. La struttura San Raffaele ha promosso ricorso al TAR Lazio, esitato nella sentenza n. 9519 del 2018, appellata davanti al Consiglio di Stato, confermata dalla pronuncia 4567 del 2019. Nel frattempo la San Raffaele SpA ha richiesto alla Regione il riesame in autotutela dell'istanza di revoca, anch'esso esitato nella nota di conclusione del procedimento del 4 ottobre 2013 con diniego. Detta nota, impugnata davanti al TAR Lazio, ha dato luogo ad una pronuncia di condanna dell'amministrazione con sentenza n. 3017 del 2014, che ha demandato all'amministrazione una nuova e compiuta istruttoria funzionale a verificare se la struttura potesse continuare ad operare in regime privatistico. L'istruttoria compiuta nel 2015 è stata dichiarata nulla, tuttavia, rinnovata dal commissario *ad acta,* ha confermato che non erano venute meno le motivazioni che avevano condotto all'adozione del provvedimento precedente. Nel merito delle rinnovate istruttorie si è poi pronunciato dapprima il TAR Lazio, con sentenza n. 9699 2018, e poi il Consiglio di Stato, a conferma del primo grado, con sentenza n. 4457 del 2019. La Regione ha sottolineato gli aspetti rilevanti della sentenza del Consiglio di Stato e come il commissario ha osservato, sebbene la struttura ha ottenuto tre certificati di agibilità dal Comune di Velletri, che coprirebbero tutte le parti in cui vengono effettuate le attività sanitarie, si deve tenere presente che il certificato di agibilità riguarda la salubrità dell'edificio. Inoltre i ricorsi promossi dall'odierno appellante avverso ai sei dinieghi opposti dal Comune di Velletri alle corrispondenti domande in sanatoria attinenti alla struttura di Velletri risultano definiti con decreti di perenzione incardinati davanti al TAR Lazio. Il diniego delle domande in sanatoria, divenuto definitivo a seguito dei decreti di perenzione, conferma l'insanabilità sul piano edilizio delle modificazioni strutturali intervenute nella struttura di Velletri dal 25 gennaio 2001. Da ultimo, la Regione Lazio ha sottolineato che la Corte di cassazione, con ordinanza n. n. 1603 del 19 gennaio 2022, si è pronunciata sul ricorso per cessazione presentato dalla San Raffaele SpA attraverso sentenze del Consiglio di Stato dichiarandolo inammissibile. Tuttavia, in considerazione - come diceva l'interrogante - del rilievo che la situazione in essere riveste in ambito territoriale nell'interesse dei cittadini, soprattutto anche per quanto riguarda i livelli occupazionali, esprimo tutta la mia disponibilità ad approfondire la disamina anche con la Regione, nel rispetto delle competenze della Regione stessa e di tutte le decisioni

La legge successiva di proroga dei termini del 2022 ha dato disponibilità a utilizzare le risorse non utilizzate dalle Regioni per abbattere le liste d'attesa. Tuttavia, il 33 per cento di queste risorse che erano state finalizzate, circa 165 milioni, non sono state utilizzate per tale scopo. Alcune Regioni hanno investito solo percentuali marginali rispetto a quanto a disposizione; altre a mala pena un terzo dei fondi stanziati. Bisogna, quindi, agire prontamente ed attivamente per la riduzione di queste liste d'attesa. È necessario intervenire in modo decisivo, con nuove regole di ingaggio degli erogatori, agendo in prevenzione e appropriatezza in tutta

dell'emergenza urgenza, il recupero dei tempi delle liste d'attesa, garantendo una prima risposta efficace sul territorio, seguita dal consulto specialistico, nell'ottica di decongestionamento dei pronto soccorsi. In proposito, anche dall'analisi del Rapporto civico sulla salute 2023 di Cittadinanzattiva, emerge che, terminata l'emergenza pandemica, i cittadini si trovano a fare i conti più di prima con le conseguenze di scelte improvvide che durano da decenni; scelte che, come ho già avuto modo di evidenziare, hanno ottenuto un solo e unico effetto: un Sistema sanitario nazionale ingolfato, un serbatoio che perde, nel quale si è sempre e solo voluto aggiungere acqua, senza riparare le falle strutturali. Le liste d'attesa non sono altro che il sintomo di un sistema da ripensare. Da ripensare è l'architettura complessiva dell'offerta sanitaria, con il potenziamento della medicina territoriale. Sono allo studio proposte concrete per l'implementazione del sistema disegnato dal decreto interministeriale del 23 maggio 2022, n. 77, accompagnato da sistemi di telemedicina e di supporto specialistico diagnostico integrato per soddisfare al meglio i bisogni degli assistiti, contrastando soprattutto gli accessi inappropriati al pronto soccorso. Accanto a questo, è altrettanto necessaria una revisione del modello di assistenza ospedaliera Venendo specificatamente all'esame di come le Regioni e le Province autonome abbiano utilizzato i fondi destinati al recupero sui ritardi accumulati nelle liste di attesa, devo premettere che il Ministero della salute ha condotto un monitoraggio sistematico dello stato di avanzamento delle attività di recupero, articolato per trimestri e prolungatosi fino alla fine del 2022. L'esito di questo monitoraggio effettivamente evidenziato, da parte degli enti territoriali, il mancato utilizzo dell'intera quota dei finanziamenti stanziati. Va precisato, tuttavia, che le quote di finanziamento non utilizzate non sono state utilizzate per per altro scopo. Il decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198, ha introdotto specifiche misure volte a favorire il recupero delle liste d'attesa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e le prestazioni ospedaliere. In particolare, è prevista la possibilità per Regioni e Province autonome, di rendere disponibile le risorse correnti, già previste nella legge di bilancio del 2021, non utilizzate al 31 dicembre 2022. Al fine di supportare le Regioni e le Province autonome nell'attuazione di quanto disposto con il summenzionato decreto legge del 2022, il Ministero ha diramato uno specifico atto di indirizzo per dare indicazioni specifiche sulle attività di recupero delle prestazioni ambulatoriali, *screening* e ricovero ospedaliero, per ridurre le liste d'attesa garantendo, nel contempo, il prosieguo delle attività di monitoraggio e supporto fornito al Ministero della Salute da Agenas. Confermo, quindi, l'intenzione di verificare ancora meglio come siano stati spesi i fondi straordinari stanziati per le liste d'attesa. Accolgo con favore le puntualizzazioni dei senatori della Lega, che ripercorrono diverse misure che stiamo sviluppando proprio nella direzione di una vera riorganizzazione della filiera della medicina territoriale e dell'emergenza-urgenza. Fatemi sottolineare che la situazione delle liste d'attesa dimostra che i fondi servono, ma ciò che soprattutto serve è saperli spendere. Il Ministero non mancherà nei controlli, ma occorre maggiore responsabilità da parte di molte Regioni nei moltiplicare gli sforzi per garantire il fondamentale diritto alla salute.

dei livelli essenziali delle prestazioni, cioè l'organo di supporto alla riforma sull'autonomia differenziata. Il 4 luglio, come sappiamo, gli ex presidenti della Corte costituzionale Amato e Gallo, l'ex presidente del Consiglio di Stato Pajno e l'ex ministro Bassanini hanno deciso di dimettersi perché, a loro dire, non ci sono più le condizioni per la partecipazione ai lavori del comitato. La ragione principale sarebbe da ricercarsi nella contraddizione tra la legge di bilancio 2023 e alcune disposizioni successive. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma infatti impone che, prima dell'attribuzione di nuovi specifici compiti alle Regioni, vengano determinati tutti i livelli essenziali delle prestazioni relativi all'esercizio dei diritti. Ma essendo le risorse disponibili definite dai vincoli di bilancio, è evidente che la determinazione dei LEP richiederà una valutazione complessiva di ciò che il Paese è effettivamente in grado di finanziare. Ciò peraltro non può essere fatto nemmeno materia per materia, perché ci si ritroverebbe nella condizione di non poter finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio dei diritti nelle materie lasciate alla fine. Non viene inoltre condiviso il ricorso alla spesa storica, che cristallizza le diseguaglianze territoriali, e si critica anche la devoluzione al sottogruppo della individuazione dei LEP nelle materie non ricomprese nel perimetro dell'articolo 116 della Costituzione. Come per gli altri LEP, il risultato sarà quello di una sola ricognizione di quelli già rinvenibili a legislazione vigente. Sarebbe stato invece utile proporre alla cabina di regia, e poi alla valutazione del Parlamento con riserva di legge, i nuovi LEP necessari per assicurare il superamento delle diseguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali. Vi sono materie, come sappiamo, nelle quali il legislatore non ha determinato i livelli essenziali delle prestazioni o lo ha fatto in modo parziale. Quindi considerando i LEP come un argomento decisivo della riforma, visto che il testo prevede che il trasferimento di competenze alle Regioni possa avvenire soltanto dietro la determinazione dei fabbisogni e dei costi *standard* effettuata dal comitato, considerando anche i rilievi di incostituzionalità che spesso sono stati sollevati nelle audizioni in 1a Commissione, considerato il rischio di aggravare le differenze territoriali, peraltro privando il Parlamento delle competenze in materia dell'allocazione delle risorse necessarie per garantire i LEP e ritenendo invece il mio Gruppo che il Parlamento possa e debba definire alcuni limiti alla negoziazione delle intese, come per esempio le norme sull'istruzione, io le chiedo se non ritenga opportuno un ripensamento su questo provvedimento e la sospensione del suo esame. Signor Presidente, in premessa ritengo necessario precisare che il comitato tecnico scientifico per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è un organismo di supporto tecnico per le attività della cabina di regia disciplinata dalla legge di bilancio per il 2023. È mia intenzione, in considerazione della natura tecnica del CLEP, di cui fanno parte 58 qualificatissimi rappresentanti delle istituzioni, esperti e accademici di varia formazione e area culturale, evitare che il medesimo CLEP sia coinvolto nel confronto politico. È necessario, proprio per le alte finalità perseguite (l'istruttoria per la determinazione dei LEP), che esso svolga la propria attività al riparo da impropri condizionamenti esterni. Quanto al quesito posto dall'interrogante, osservo che esso è diretto a produrre la sospensione dell'esame del disegno di legge n. 615. Altri sono gli strumenti previsti dal Regolamento del Senato per giungere a tale risultato, dal Governo ovviamente non auspicato, e non certo gli strumenti del sindacato ispettivo. Nel merito, devo ribadire che, diversamente da quanto sostenuto - senza in realtà addurre argomenti - dall'interrogazione, non sussiste alcuna contraddizione nelle disposizioni della legge di bilancio per il 2023 che invece legano indissolubilmente ed espressamente il processo di emanazione dei LEP alle materie interessate dall'autonomia differenziata. Sono inoltre immotivate le critiche relative all'istituzione di un ulteriore sottogruppo, chiamato a istruire la determinazione dei LEP in tutte le ulteriori materie. Al contrario, il CLEP ha accolto la richiesta dei quattro firmatari della lettera. Il sottogruppo, diversamente da quanto ivi sostenuto, non sarebbe chiamato a svolgere una mera opera di ricognizione dei LEP già rinvenibili nella legislazione esistente, ma, al pari degli altri sottogruppi, dovrebbe proporre, nel caso, anche nuovi LEP nell'ambito delle funzioni esistenti, necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali. I diritti civili e sociali sulla base delle chiare riserve contenute nella prima parte della Costituzione, sono stabiliti dalla legge, così come è la legge che disciplina l'attribuzione all'esercizio delle funzioni pubbliche. È sempre in base alla legge che saranno determinati i LEP con i decreti del Presidente del Consiglio. Il ricorso ai decreti agevola il tempestivo adeguamento nel tempo dei LEP alle mutate esigenze e condizioni, non ultime quelle derivanti dal mutato quadro tecnico scientifico. Il Governo non è certo insensibile alle molteplici questioni poste nel corso del dibattito parlamentare e delle audizioni e farà proprie alcune proposte emendative di carattere migliorativo dei contenuti del disegno di legge. È certo però che non è consentito alla legge ordinaria, come vorrebbe l'interrogante, porre limiti preventivi ai contenuti delle intese, relativi a materie specificatamente indicate nella Costituzione. ad occuparsene, quando esaminerà le singole ipotesi, con gli atti di indirizzo prima e il voto finale a maggioranza assoluta poi.

nei prossimi giorni potranno effettivamente cambiare natura in maniera significativa a questo provvedimento. Lei conosce la nostra posizione, la grande perplessità

un grande elemento di perplessità trasversale attorno a questa riforma. Soprattutto, Ministro, c'è la grande preoccupazione che questa sua riforma possa aggravare la diseguaglianza sociale e la diseguaglianza territoriale, che sono già oggi purtroppo la cifra più significativa di questo Paese. Io penso che lei abbia visto, come me, gli ultimi dati che sono usciti ieri sulla scuola, che sono drammatici perché parlano di un divario territoriale tra le scuole del Nord e le scuole del Sud, che comincia a manifestarsi addirittura già nella scuola primaria, con -15 per cento punti di divario a sfavore del Mezzogiorno al termine del primo ciclo della scuola secondaria, e -23 per cento al termine del secondo ciclo. ciclo. In un Paese purtroppo così segnato dal divario territoriale bisognerebbe investire sulla coesione territoriale, che penso sarebbe peraltro l'unico modo per mettere il Paese in una condizione migliore sull'intero panorama europeo. Lo dico con una battuta perché non ho il tempo: penso che questa riforma rischia di essere drammatica per il Sud, ma anche una riforma profondamente sbagliata per il Nord. È tutto il Paese che ne uscirà indebolito. Spero davvero, finendo come ho iniziato, che gli emendamenti possano cambiarne significativamente il segno. In ogni caso, la ringrazio della risposta.

hanno rassegnato le dimissioni dal Comitato tecnico per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, presieduto dal professor Sabino Cassese. Lo hanno fatto con una lettera nella quale avanzano molteplici e seri dubbi sulla conformità alla Costituzione del disegno di legge n. 615 che stiamo discutendo in Commissione affari costituzionali e che porta la sua prima firma. In particolare avanzano seri e molteplici dubbi sul percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, che tale disegno di legge prefigura. La principale questione che viene sollevata nella lettera riguarda il rapporto tra articolo 116, terzo comma, e articoli 117, lettera *m)*, e 119. È possibile e costituzionalmente legittimo procedere all'attribuzione di nuovi e specifici compiti e funzioni ad alcune Regioni, con le corrispondenti risorse finanziarie, senza aver previamente determinato e concretamente attuato tutti i i livelli essenziali delle prestazioni attinenti all'esercizio dei diritti civili e sociali ed aver previamente definito il loro finanziamento secondo i principi dell'articolo 119 della Costituzione? Ecco, ad avviso dei quattro illustri giuristi, ciò non dovrebbe avvenire. Una corretta lettura del Titolo V dovrebbe escludere una simile eventualità perché prima occorre garantire le condizioni essenziali dell'uniformità, prima occorre superare i divari territoriali territoriali e garantire a tutti i cittadini, ovunque risiedano, il pieno godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali e, solo dopo, valutare se e per quali specifiche funzioni e compiti è ragionevole prevedere differenziazioni e dunque forme e condizioni particolari di autonomia a una o più Regioni. Siccome però le risorse di cui il nostro Paese dispone sono necessariamente limitate, perché ciò avvenga occorre che il Comitato tecnico proceda alla determinazione di tutti i livelli essenziali delle prestazioni relative all'esercizio dei diritti civili e naturalmente vi provveda superando il criterio della spesa storica, che riflette e consolida le disuguaglianze territoriali esistenti, in modo da consentire al Parlamento di fare una valutazione complessiva delle risorse che sono necessarie per finanziare tali LEP e decidere di conseguenza, nel rispetto della Costituzione, priorità e grado della loro attuazione. Ma se il comitato tecnico procederà invece alla determinazione dei soli livelli essenziali relativi alle materie potenzialmente oggetto di autonomia differenziata, come potranno il legislatore e lo stesso Governo scongiurare il rischio che alla fine manchino le risorse per finanziare tutti i LEP necessari ad assicurare l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato? E come potrà, quindi, garantire la previa, concreta ed effettiva attuazione dell'articolo 117 della Costituzione? Le chiediamo dunque, signor Ministro, di rispondere alle questioni e ai dubbi di legittimità sollevati nella lettera. Avremmo voluto interloquire e ci sembra ragionevole che ciò avvenga anche con il comitato tecnico, ma in ogni caso

superando i rischi di legittimità costituzionale che sono stati evidenziati nella lettera che ho richiamato.

quindi che si debba ribadire e precisare che il CLEP è stato istituito con un DPCM del 23 marzo 2023, quale organismo di supporto tecnico per l'attività della cabina di regia, disciplinata dalla legge di bilancio. È vero che in quattro hanno hanno presentato una dichiarazione di non partecipazione ai lavori, ma ce ne sono altri 58, altrettanto qualificati, che intendono procedere per la strada individuata, che andrò a ripetere, perché è sovrapponibile a quella che è stata indicata dai quattro Nel merito devo precisare che mi sono meravigliato nell'apprendere che è stata data pubblicità al contenuto di una lettera, con cui i quattro firmatari mi avevano rappresentato di essere «costretti «costretti a prendere atto che non ci sono le condizioni per una nostra partecipazione ai lavori del CLEP». Nel merito devo precisare che fin dall'inizio era stato chiarito e condiviso per iscritto, con i quattro firmatari, il perimetro dell'attività del CLEP, in attuazione delle disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto dal DPCM. In un momento successivo, i quattro hanno rappresentato insieme al CLEP, oltre che al sottoscritto, l'esigenza di estendere tale perimetro anche alle altre materie, adducendo argomenti non privi di rilievo, indicati nella loro lettera. Proprio per questo il CLEP ha accolto la richiesta di estendere l'istruttoria ad ulteriori materie e ha convenuto di istituire a tal fine un ulteriore sottogruppo. Quest'ultimo, a sua volta, diversamente da quanto posto in evidenza nella lettera, non sarebbe chiamato a svolgere una mera opera di ricognizione dei LEP già rinvenibili nella legislazione esistente, ma al pari degli altri sottogruppi dovrebbe proporre, nel caso, anche nuovi LEP nell'ambito delle funzioni esistenti, necessari per assicurare effettivamente il superamento delle disuguaglianze territoriali nell'esercizio dei diritti civili e sociali. Quanto alla pregiudizialità relativa all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, gli stessi interroganti, riportando un passo della lettera, pongono in evidenza che il solo limite di rango costituzionale è dato dal rispetto dei princìpi dell'articolo 119, nessuno dei quali è posto minimamente a repentaglio nell'attuazione dell'autonomia differenziata, né tantomeno dal disegno di legge n. 615. Non posso che ribadire che i dubbi di legittimità prospettati sono privi di fondamento e che proprio il sottoscritto e il Governo intero si stanno facendo carico, finalmente, del processo attuativo dei LEP, a distanza di oltre ventuno anni dall'entrata in vigore del Titolo V. Concludo con due valutazioni politiche. La prima è che uno dei firmatari di questa lettera era Presidente del Consiglio quando fu approvata la modifica del Titolo V. Gli interroganti appartengono all'area politica che fu promotrice, votò e sostenne il *referendum* rispetto alla modifica del Titolo V. Sono passati più di vent'anni e per tredici anni questa area politica è stata, con Governi politici o tecnici, al Governo. Lei ha ripetuto tante volte la parola «prima» io adesso dico «prima o poi», perché dopo questi tredici anni e ventuno anni nessuno ha fatto un passo in avanti sull'autonomia, nessuno si è mai incaricato né si è voluto dedicare alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

portata avanti da me e poi sospesa dai Governi che sono succeduti. La lettera *p)*, la definizione della funzione fondamentale, ha trovato ancora una volta contenuto nella mia riforma del federalismo fiscale. Oggi dire che dobbiamo definire tutti i LEP prima di poter procedere significa solo buttare la palla in tribuna, disconoscere quei troppo pochi livelli essenziali già definiti ad oggi e quando oggi uno dice di volere tutto di fatto non vuole dire niente e tra vent'anni saremo ancora qui a parlare di definizione di livelli essenziali che lo Stato ha il dovere di definire e dei diritti civili e sociali che il cittadino ha diritto di vedersi garantiti.

la sua risposta ci lascia amareggiati, ma direi addirittura sgomenti rispetto alle esperienze e al profilo che lei stesso, Ministro, ha all'interno di quest'Aula e del percorso istituzionale e parlamentare di questo Paese. Paese. Nella risposta al collega De Cristofaro - e mi voglio augurare non facesse riferimento al ruolo del Parlamento - ha parlato di impropri condizionamenti esterni rispetto al lavoro di un comitato tecnico. Le vorrei semplicemente ricordare con pacatezza

L'unico depositario, quindi, della scelta dei livelli essenziali delle prestazioni è e resta il Parlamento, al di là delle valutazioni di questo Governo. anche in chiacchiere informali, al fatto che in qualche modo queste erano scelte tecniche. Ebbene queste scelte e questi quattro autorevoli giuristi la cui appartenenza penso non faccia velo però alla loro competenza, al merito delle loro argomentazioni, merito delle argomentazioni che la vostra stessa decisione, la scelta del comitato tecnico di istituire un sottogruppo, che evidentemente riconosce. I firmatari di quella lettera hanno detto che la scelta non li convince e non perché pensino che quel sottogruppo non sia dedicato esattamente alla ricognizione, che quindi voi avete riconosciuto come essenziale. Al di là dello sproloquio sul fatto che poi questi livelli essenziali, tutti o non tutti, vadano evidentemente individuati, individuati, voi stessi riconoscete che è necessario, perché avete individuato un sottogruppo che deve definire anche quelli non oggetto della devoluzione. Ma quel sottogruppo - hanno detto i quattro firmatari - non avrà i tempi necessari, se proprio la vogliamo fare sul serio quella individuazione, per lavorare e arrivare alla definizione, quindi hanno detto che sostanzialmente si sta facendo un'operazione di facciata. Adesso capisco che ci sono bandierine ideologiche per parti politiche, lo comprendiamo, siamo tutti quanti navigati, ma attenzione a giocare queste

una forza politica, ma anche l'intera maggioranza se ne assume la responsabilità di fronte alle eventuali conseguenze che ci saranno nel corso degli anni. Attenzione a dire, e in qualche modo a rivendicare, rivoluzioni importanti e necessarie attese da anni: noi le vorremmo fare, ma con serietà e rigore e, soprattutto, perseguendo gli obiettivi che si dice di voler perseguire.